per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1, a firma dei senatori Lumia, Pagnoncelli, Romano, Cervellini e Scavone, e sono state contestualmente ritirate tutte le mozioni ad eccezione della mozione

in questa discussione, che ha visto numerosi e precisi interventi, si è sviluppato un confronto che ha messo in condizioni anche noi, del

perché il dato che emerge non può essere iscritto nelle difficoltà rituali: siamo di fronte ad un vero e proprio dramma,

di vita di tantissimi, centinaia di migliaia, milioni di donne e di uomini italiani perduti fisicamente dentro l'atto dell'azzardo. Perduti in termini di qualità di una vita non più riconosciuta,

questa situazione drammatica che coinvolge non a caso i ceti più deboli, più esposti. Dal punto di vista generazionale

Credo che è su questa solitudine sociale che noi dobbiamo assolutamente agire. Il punto è avere tutti gli strumenti per intervenire e adottare

hanno visto innalzare il picco della piaga del gioco d'azzardo. È in questo senso che ci dobbiamo muovere e lì possiamo cominciare a trovare il bandolo della

una delle forme più organizzate e capillari all'interno del nostro Paese. Se penso a una città come Roma, dalle zone più centrali fino a quelle più periferiche, le sale giochi, le macchinette, questi luoghi organizzati sono forse la presenza più diffusa:

e colleghi, presentarci in Aula con questo lavoro di sintesi sulle mozioni che i vari Gruppi hanno presentato su problema così drammatico che investe tutti noi è la maniera migliore per ricominciare e per parlare di un Paese che troppo spesso ha avuto punte di ipocrisia e di disordine che sono purtroppo caratteristiche della nostra latitudine.

la chiusura del casinò di Taormina, che drammaticamente trasformò una delle perle del Mediterraneo, facendola decadere

che ha previsto a tutela dei cittadini più fragili e più esposti una forma di attenzione e di prevenzione che però non è stata

delle autorizzazioni. Già nel 2011 era stato previsto un concerto tra i Monopoli di Stato ed il Ministero della salute per l'emanazione di un decreto interdirigenziale che normasse, tutelasse e seguisse complessivamente l'evoluzione di questo tragico spaccato che investe la gran parte della popolazione del nostro Paese;

un inserimento stabile nel mondo del lavoro inducono questa fascia di popolazione, la più fragile e la più esposta, a rifugiarsi

forti di una normativa che ha consentito, attraverso un sistema delle concessioni a distanza, arricchimenti anche

pressante che il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, aderendo al lavoro comune di sintesi delle mozioni, chiede di impegnare il Governo a far bene, a far seriamente, a tutelare i nostri giovani,

La questione è molto semplice. Non occorrono altri dati, ma ne leggerò comunque qualcuno: 100 miliardi di euro di fatturato, 4 per cento del PIL nazionale, terza industria nazionale, 8 miliardi di euro di tasse; il 12 per cento della spesa delle famiglie finisce nel gioco d'azzardo; 400.000 *slot machine*; 6.181 locali ed agenzie autorizzate; 15 milioni di giocatori abituali; 3 milioni a rischio patologico,

Questi sono i numeri del gioco lecito, a cui va aggiunta la sfera dell'ignoto che sta nel sommerso dell'illecito. E allora, a fronte di questo, abbiamo ascoltato il territorio. Questo non è altro che il manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo. Proprio qualche settimana fa, in quest'Aula, è stato approvato nel decreto del fare un provvedimento ai sindaci, su loro esplicita richiesta, di rimanere seduti nei banchi del Parlamento: lo hanno voluto, lo hanno preteso. Vorrei vedere oggi i sindaci esprimersi in coerenza con questo manifesto, non in coerenza con gli interessi di chi, invece, sta dietro al gioco d'azzardo e, quasi sempre, è malavita, malaffare, o comunque cosa slegata dall' interesse dalle famiglie. Anche qui vedremo la coerenza o l'ipocrisia. Ma diciamo anche una cosa. Noi ci siamo mossi anzitempo, perché, ascoltando i territori, abbiamo presentato una mozione, il 29 maggio, chiedendo una moratoria al Governo, chiedendo innanzitutto di frenare la diffusione delle macchinette e delle *slot machine*, che da sole producono circa la metà di quello che il Governo incassa e che mette poi nel proprio bilancio: 7 miliardi di euro. In seguito abbiamo visto presentare altre mozioni che ci fosse veramente un'intenzione di porre freno a questo degrado, che non è solo morale, ma è soprattutto economico - ripeto - e che sta mettendo in grave difficoltà le nostre famiglie. Abbiamo visto presentare mozioni da parte di tutti i Gruppi e abbiamo assistito ieri a rituali che portano poi, o dovrebbero portare, a sintesi di buonsenso. Ci è stato proposto di far confluire la nostra mozione in una proposta di maggioranza; vi abbiamo inserito all'interno le nostre proposte di moratoria, ma subito ci siamo accorti che qualcosa non quadrava. E anche qui chiederei coerenza da parte di quei senatori che si sono detti d'accordo nel sostenere una moratoria per nuove licenze: nel risistemare quello che già esiste prima di concedere nuove licenze; chiederei di mantenere fede a quello che si è detto ieri e di non subire poi la pressione di chi ricatta il Governo per dire che, senza nuove licenze, non verrà pagata la sanatoria che tiene in piedi il decreto IMU. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Questo è quello che deve essere detto e quello che ciascuno deve avere presente quando si andrà poi a votare. Altrimenti gli interessi del Paese finiscono proprio nascosti dietro quell'ipocrisia che si vuole smascherare. Questo provvedimento per il Governo è necessario; mantenere i proventi del gioco d'azzardo è necessario per garantire la tenuta dei conti dello Stato. Ed è una gravissima ipocrisia. Agli italiani bisogna chiedere nuovi sacrifici, ma non sacrifici che siano mascherati dal dal lucro fatto sulle tasche dei meno abbienti, perché ricordiamo che ciò di cui stiamo parlando non è il gioco d'azzardo, che esiste da quando esiste l'uomo. Stiamo parlando di una diffusione capillare nelle famiglie, attraverso punti di gioco che si sono diffusi come funghi nei bar e in ogni luogo pubblico nel Paese. Questa è una situazione immorale che si è venuta a creare nel Paese, non in cinquant'anni, ma nel corso degli ultimi anni. A fronte di questo, chiedo anche ai senatori che siedono qui dentro e che hanno votato quelle leggi che consentono questo stupro del territorio di porvi fine e di porvi rimedio. Si può ancora fare.

è una valutazione che viene condivisa da chi, sul territorio, (il terzo settore) ha poi a che fare con coloro che sono danneggiati dal gioco d'azzardo patologico. A fronte di questo chiediamo quindi un impegno. Ovviamente noi manterremo la nostra mozione. Chiediamo il buon senso dei senatori e chiediamo ai Gruppi di essere coerenti con la loro missione di rappresentanti del popolo. Non chiediamo invece ai senatori di essere sottomessi a quel ricatto che induce oggi il Governo a non accettare la moratoria. Chiediamo al Senato di far vedere che la politica può ancora avere un significato nel Paese e che non soggiace agli interessi economici che, come nel caso del gioco d'azzardo, che ha causato quell'enorme buco e quell'enorme mancato introito, si sono visti poi ricollegati alla mafia e a tutto quello che è il malaffare e al malcostume che vi stanno dietro. Su questo si vedrà la vera coerenza di questo Senato e dei senatori che vi siedono, con il mandato popolare ricevuto. Qui si vedrà l'ipocrisia, e noi saremo coerenti con il mandato che abbiamo ricevuto dalla nostra gente, perché difendiamo gli interessi dei cittadini, a partire dalle famiglie più deboli.

l'ordine del giorno e le mozioni su cui oggi abbiamo la responsabilità di pronunciarci pongono questioni cruciali per comprendere il valore che attribuiamo alla funzione dello Stato. Nessuno immagina uno Stato etico, che imponga costumi e modelli di vita, ma neppure, al contrario, possiamo accettare che lo Stato divenga un biscazziere, che non si ponga il problema della difesa dei più deboli, che ignori la sua funzione educativa. L'incidenza del fenomeno del gioco d'azzardo,

Tale documento, discusso in quest'Aula nell'ottobre del 2011, concludeva: «Sin d'ora appare, comunque, in tutta evidenza come il settore del "gioco" costituisca il punto d'incontro di plurime, gravi distorsioni dell'assetto socioeconomico quali, in particolare, l'esposizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; l'interesse del crimine organizzato; la vocazione "truffaldina" di taluni concessionari che operano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri fenomeni criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la sottrazione di ingenti risorse destinate all'erario. Il paradosso più evidente si ravvisa nel fatto che lo Stato, per un verso, recuperi risorse finanziarie attraverso la diffusa "tassazione indiretta" dei redditi e, per altro verso, sia esso stesso sistematicamente "depredato" dalla contestuale esistenza di meccanismi truffaldini di gioco non censito». La diffusione estesa sul territorio delle più fantasiose forme di tassazione indiretta, derivante dal cosiddetto gratta e vinci, dal lotto e dalle sue varianti, da *slot machine* e sale bingo, dal gioco via Internet, dal *videopoker*, in verità alimentano la malattia del gioco,

a fronte di una crisi economica che presenta fenomeni degenerativi, che mette a repentaglio la tenuta dei redditi delle famiglie, ma soprattutto la loro speranza di queste nel futuro e che incentiva quindi, nei soggetti che maggiormente vivono la crisi e avvertono la disperazione del momento, il desiderio di trovare una facile via d'uscita, che mai lo Stato dovrebbe fornire. abbiamo il dovere di far sì che i nostri concittadini scommettano, ma la scommessa deve essere per il bene delle persone, sul futuro, per il lavoro, la famiglia,

e con un cinismo spesso inaccettabile, stiamo incentivando la scommessa sul nulla, che produce impoverimento, frustrazione, cancellazione del futuro. Le tante tragedie che si sono consumate in questi anni a causa del gioco d'azzardo, l'ansia spesso nascosta (un fenomeno che in molti casi non compare sulle cronache dei giornali, se non quando arriva al livello di tragedia, ma che è presente nella vita delle famiglie) che tanti vivono nel sogno di una vincita, sprecando risorse molte volte indispensabili per una vita dignitosa, ci impegnano a cambiare. Signor Presidente, colleghi, Scelta Civica voterà oggi l'ordine del giorno proposto, ma contestualmente invita con forza il Governo ad assumere tutte quelle decisioni rigorosamente conseguenti

quelle che ne sono le conseguenze, cioè la necessità di reperire risorse sostitutive di quello che riteniamo un ingiusto guadagno da parte dello Stato. salutiamo in tribuna il sindaco di Zagabria, Milan Bandȋc, che sta seguendo i nostri lavori, cui diamo il benvenuto qui, al Senato della Repubblica italiana.

Signor Presidente, distinti colleghi, non giriamo attorno alle cose: lo Stato è sotto processo morale per aver incitato al gioco i cittadini nella illusione di fare cassa sulle sofferenze ed è chiamato ad un riscatto pronto e pieno. Il vice ministro Bubbico si è impegnato in questo senso, a parole, e lo stesso ministro Zanonato ha mostrato disponibilità. Vedremo. Abbiamo assistito a troppe inerzie e promessa da marinaio, fino ad oggi. Già la legge di stabilità 2010 per l'anno 2011 prevedeva l'emanazione di un decreto per contrastare il gioco d'azzardo patologico. Il 29 giugno 2011 il Senato approvò la mozione n. 441 che impegnava il Governo a normare la pubblicità e introdurre messaggi deterrenti, tessere elettroniche a tutela dei più giovani e a destinare quote delle maggiori entrate ad interventi di prevenzione e cura delle forme compulsive da gioco. Tanto la legge quanto la mozione rimasero lettera morta. Il 1° agosto 2012 intervenne il TAR del Lazio accogliendo il ricorso presentato da Codacons e ordinò di adottare, entro 60 giorni, il decreto di cui sopra. Così siamo arrivati al cosiddetto decreto Balduzzi, che istituiva finalmente l'ingresso nei livelli essenziali di assistenza

Da notare che quel decreto si intitolava «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute». Si ammetteva implicitamente che questa industria è dannosa allo sviluppo del Paese. Dunque, l'ora non è più rinviabile. Non è il momento di mezze misure, anche perché la politica deve finalmente fare un passo avanti recuperare la credibilità persa nella matassa dei conflitti di interesse. Ricordo che tra il 2004 e il 2006 i dieci principali gestori del mercato delle *slot machine* evasero ed elusero sistematicamente i controlli fiscali tenendo scollegati gli apparecchi dai sistemi di rilevamento degli incassi. Il colonnello Rapetto, della Guardia di finanza, riuscì a scoprire e documentare l'entità delle violazioni: 98 miliardi di euro, 50 euro per ogni ora di mancato collegamento. dell'intero debito delle amministrazioni pubbliche verso le imprese private. Per abolire l'IMU sulla prima casa basterebbero quattro Aggiungo che Giorgio Tino, parente dell'ex ministro Antonio Maccanico, e Antonio Tagliaferri, rispettivamente direttore generale e direttore del settore giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per le gravi omissioni nei controlli di loro competenza furono condannati a risarcire 16 e 8 milioni di euro Il ministro Tremonti volle una commissione, che ridimensionò la sanzione di oltre cento volte, da 98 miliardi a 800 milioni. A presiederla il ragioniere generale dello Stato, Andrea Monorchio, che fatalmente era anche presidente di una delle società multate. La Corte dei conti decise poi di applicare un criterio diverso, basandosi sul danno presunto per l'Erario e rideterminò la sanzione, portandola a 2,5 miliardi. Ma è come dire che, se io passo con il rosso, mi appello al danno presunto e, se non ho prodotto un incidente, chiedo che la multa mi venga ricalcolata o addirittura azzerata. Anche ai dirigenti dei Monopoli di Stato Tino e Tagliaferri la sanzione fu ridotta, adducendo il fatto che in fondo tutte le società avevano evaso. Ma è come dire che, se un vigile si distrae controllando il traffico, viene sanzionato, ma se si addormenta del tutto, la sanzione viene ridotta del 70 Le concessioni, ricordiamolo, non furono revocate, anzi le società ne ottennero di nuove e più redditizie. Giorgio Tino non fu licenziato e nel 2009 divenne addirittura vice presidente di Equitalia e presidente di Equitalia Veneto. Antonio Tagliaferri rimase al suo posto e nel 2012 venne pure riconfermato dal Governo Monti. Il colonnello Rapetto, invece, si trovò costretto alle dimissioni. Arriviamo alla nascita di questo Governo. Il 28 aprile 2013, durante il giuramento, un uomo rovinato finanziariamente e psicologicamente dal gioco d'azzardo spara e colpisce davanti a Palazzo Chigi il brigadiere Giuseppe Giangrande e l'appuntato Francesco Negri, due servitori dello Stato, quello Stato che per mano dei Governi staffetta di centro-destra e centro-sinistra ha permesso di portare macchinette mangia soldi fin dentro i circoli sportivi e parrocchiali. Il 22 maggio riportai in Aula la denuncia di Matteo Iori sui rapporti tra politica e industria del gioco d'azzardo, che finanziava generosamente UDC, Margherita, Democratici di Sinistra, MPA di Lombardo, candidati candidati di spicco come Gianni Alemanno e Amedeo Laboccetta, fondazioni come "VeDrò", riferibile al presidente del Consiglio Letta, a sei Ministri del suo Governo, al suo vice, Alfano, o a politici come Matteo Renzi... che assumeva o affidava cariche ad ex ministri come Vincenzo Scotti e Augusto Fantozzi o all'onorevole Francesco Tolotti. Per non dire dei politici entrati in affari nel settore, come Marina Berlusconi, i figli di Clemente Mastella e Marcello Dell'Utri. Io invitavo a tagliare di netto queste relazioni, legali, ma politicamente pesantissime, per sgomberare il dibattito a venire da questi dubbi. Invece il Governo Letta, alla vigilia di questi atti di indirizzo, anziché fugare i dubbi, conferma di esserci dentro con mani e piedi. Ha infatti inserito fresco fresco un condono nel decreto IMU proprio per le società

Letta potrebbe, in qualche modo, finanziare la soddisfazione di "*Mister* B" e le sue pretese sull'IMU, mentre Corallo, dopo 14 mesi di latitanza, potrà tornare alle Antille con duecento milioni di euro. Ma non è tutto, perché queste società sanno di poter ottenere di più. Se questo è lo stato di scacco del Governo potranno rinegoziare questa sanzione residua chiedendo magari il prolungamento delle concessioni in atto oppure nuove concessioni o chissà che altro. Noi su questo vogliamo vederci chiaro, perciò abbiamo inserito un punto irrinunciabile nella nostra mozione, ossia che questo condono venga stralciato nel momento in cui il decreto approderà in Aula e che si dia corso a tutte le azioni per esigere integralmente il pagamento delle sanzioni, nonché la rimozione immediata (misura che

dunque anche gli altri partiti, e ogni singolo senatore, a mettersi una mano sulla coscienza e a valutare punto per punto le nostre proposte, per le quali chiederemo la votazione per parti separate. *(Applausi

sino a dieci anni fa le scommesse in Italia erano esclusivamente nelle mani della criminalità organizzata. Le *slot machine* non erano *online* e il giro d'affari, pur notevole, era comunque contenuto. Poi lo Stato ha iniziato ad occuparsene, per regolare un settore in continua crescita, nel quale vi era da colmare un vuoto legislativo, con l'obiettivo di introdurre nuove offerte di gioco d'azzardo pubblico. Solo pochi anni fa le entrate dei giochi avevano già raggiunto la cifra di 61 miliardi di euro (pari a quasi il 4 per cento del Prodotto interno lordo). Oggi il fenomeno è cresciuto, anche grazie alla diffusione sul *web* delle videolotterie e dei minicasinò. Dal 18 luglio 20111, infatti, è possibile giocare a *poker* dal *computer* di casa. È un affare da un miliardo e e mezzo di euro al mese. Nessun controllo rigoroso sulla vera età dei giocatori, cifre da capogiro mosse con un semplice *clic*, e denari italiani che volano verso altri Paesi senza la possibilità di essere intercettati dal fisco. Fino a un paio di anni fa chi voleva giocare doveva almeno entrare in una ricevitoria. Ciò significava doversi muovere fisicamente, rispettare gli orari di apertura dei giochi e dell'attività commerciale, utilizzare denaro contante. Il controllo sui comportamenti compulsivi era sicuramente più agevole, così come era più facile accertare l'età anagrafica di chi giocava. è dunque l'esigenza immediata, se non si vuole fare una moratoria, di regolare in modo molto più rigido le nuove concessioni; di controllare in modo più incisivo il *web* e di fare non uno, ma e di fare non uno, ma 100 passi indietro su alcuni giochi che di ludico ormai non hanno proprio più nulla. È vero, tuttavia, che lo Stato è riuscito in qualche modo a frenare il gioco d'azzardo illegale. In Italia, infatti, la regolamentazione del gioco distingue in maniera netta i giochi non consentiti da quelli consentiti: per i primi viene fatto assoluto divieto di offerta da parte di chiunque; per i secondi, l'offerta è subordinata ad una apposita autorizzazione. Ma anche su questo tipo di autorizzazione è necessaria una stretta energica. La ludopatia, infatti, è ormai a tutti gli effetti una malattia sociale, e per questo motivo Regioni e Comuni hanno cominciato a emanare i propri regolamenti per arginare la diffusione del gioco d'azzardo, creando in questo modo una notevole confusione in quanto lo Stato ha una riserva stabilita dalla Costituzione in materia di regolazione del gioco pubblico. Il gioco d'azzardo va dunque inquadrato anche, e soprattutto, nell'ottica di un problema di salute, trattandosi di una vera e propria malattia sociale, tanto è vero che nella passata legislatura il ministro Balduzzi ha obbligato gli esercizi commerciali a esporre avvisi sulla malattia del gioco: una misura opportuna ma del tutto insufficiente. Le leggi nazionali ed europee sulla liberalizzazione dei mercati e sul sistema delle licenze contengono ancora, infatti, evidenti contraddizioni e lacune, lasciando troppo spazio a siti di gioco d'azzardo illegale. È dunque indifferibile un intervento più puntuale a livello normativo per rendere più efficace il sistema delle autorizzazioni, dei controlli e delle sanzioni. Anche perché, oltre all'esigenza di fronteggiare una piaga sociale, di cui si occupa l'ordine del giorno congiunto che ci apprestiamo a votare, vi è una realtà ancora più inquietante, che è quella dei giochi gestiti dalle mafie, divenuti un canale privilegiato per il riciclaggio di denaro sporco. La mozione del PdL, che poi è confluita nell'ordine del giorno unitario G1, chiedeva una cosa molto semplice, cioè che venisse data attuazione al decreto-legge n. 158 del 2012, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto per la progressiva introduzione di idonee soluzioni tecniche volte ad avvertire i giocatori dei pericoli di dipendenza dal gioco. anche perché il provvedimento in questione pone finalmente un argine severo alla diffusione dei messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche e via Internet*.* Nonostante questo, però, la situazione è addirittura peggiorata, con un autentico *boom* relativo proprio al gioco d'azzardo. Occorre dunque mettere in campo mezzi adeguati perché, nel più breve tempo possibile, possano essere approvate e attuate le disposizioni contenute nel decreto, per evitare che il fenomeno della ludopatia continui ad aumentare in modo esponenziale e per tutelare le persone più esposte al rischio, come i minori o come le vittime della crisi economica, che cercano una via di fuga nella pericolosa scorciatoia del gioco d'azzardo. Bisogna infine elaborare una strategia normativa *ad hoc* per il gioco *on line* dal *computer* di casa, che rappresenta al momento una minaccia praticamente incontrollabile.

Signor Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici, ringrazio tutte le colleghe e i colleghi che sono rientrati in Aula e che stanno partecipando a questo momento importante della vita del Parlamento. Non è la prima volta - qualcuno ricordava - che si tratta questo importantissimo e delicato argomento, forse è la prima volta che si entra nel merito e che, attraverso la discussione e la votazione di questo ordine del giorno, si prova a ottenere risultati. Naturalmente, è nelle mani del Governo e del nostro Parlamento praticare poi nel concreto e nei fatti quello che nell'ordine del giorno sosteniamo. Abbiamo lavorato nelle ultime ore e fin dalla giornata di ieri per comporre un ordine del giorno che coniugasse diverse ragioni e che addivenisse ad una sintesi tra diverse proposte. Ci siamo riusciti ed io accolgo favorevolmente anche la disponibilità del Movimento 5 Stelle, che rimane forte nella sua proposta, a votare comunque l'ordine del giorno G1 su cui tanto abbiamo lavorato. Ringrazio il senatore Lumia,

perché, con i loro interventi, hanno rafforzato una linea e un orientamento del Partito Democratico, che ha anche alle spalle l'elaborazione di proposte di legge in materia che ci auguriamo possano essere presto discusse. Hanno ragione quanti hanno sostenuto che siamo di fronte a un gravissimo problema, che non va trattato con un moralismo di facciata, ma da parlamentari, cioè come coloro che, capaci di legiferare e di orientare le azioni del Governo, provano a invertire una rotta. Non siamo più al gioco della lotteria di Capodanno o a quando, ragazzini, accompagnavamo i nostri genitori o nostro padre a giocare la schedina. Siamo a una vera e propria patologia sociale, che assume forme drammatiche e che spesso riduce persone

e fino ad assumere sembianze e dimensioni drammatiche. Il gioco d'azzardo è stato, fino ad oggi, in qualche modo riorganizzato e regolato, ma non basta.

queste entrate, per la prima volta nella storia del nostro Paese, al finanziamento della ricostruzione post terremoto. In realtà - e lo dico con amarezza - da quel canale finanziario sono arrivate solo delle briciole: voglio registrarlo in quest'Aula nel momento in cui ragioniamo su quali altre entrate e quali altre possibilità possano derivare dal canale del gioco.

della camorra, della mafia, della 'ndrangheta o della sacra corona unita. Ci vuole allora fermezza ed un gesto di responsabilità: è per questo che abbiamo condiviso un testo che non dimentica l'importanza delle entrate, ma che segna in qualche modo una svolta e

innanzitutto il richiamo alla legge Balduzzi, non è possibile che una legge dello Stato indichi la necessità di decreti del Presidente del Consiglio e di altri Ministri e che poi questi decreti non vengano adottati, lasciando sospese delle soluzioni e delle proposte già adottate. Torniamo quindi su questo, chiedendo che vengano adottati tempestivamente i decreti necessari, ai fini dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per il gioco d'azzardo patologico. Nell'ordine del giorno focalizziamo anche la problematica dei minori. assessore alle politiche sociali del mio Comune di appartenenza ho trattato numerosissimi casi di minorenni che hanno completamente perso la strada dietro al gioco patologico.

all'uso del denaro: e qui entra in gioco anche il mondo della scuola e il Ministero dell'istruzione. Ci sono poi dei punti sui quali voglio soffermarmi, perché sono importanti e innovativi, e non possono essere assolutamente considerati come ordinari. Vi sono, innanzitutto, alcune indicazioni al Governo per legiferare sul divieto della pubblicità del gioco d'azzardo, sulla necessità di elevare gli *standard* di accreditamento dei concessionari e di rafforzare il sistema della tracciabilità del denaro, nonché sulla necessità di introdurre il divieto di partecipazione a gare e procedure per il rilascio di concessioni in materia di giochi da parte di persone fisiche fisiche e giuridiche condannate per reati gravi, anche in via non definitiva, perché è lì che si creano i legami con la mafia, con la camorra e con i *clan* che purtroppo imperversano in gran parte del nostro Paese. di inasprire le pene per tutti i reati relativi al mercato dei giochi e di rafforzare i livelli investigativi delle procure e dei reparti specializzati delle forze di polizia. sindaci, che hanno bisogno di più poteri in materia di autorizzazioni e di considerare, nell'ambito di un'organizzazione generale delle proprie attività, quali e quante autorizzazioni debbano essere rilasciate nei loro Comuni. Nell'ordine del giorno chiediamo di istituire meccanismi per verificare la maggiore età del giocatore per l'accesso ai giochi *online*, che proliferano

l'allineamento dell'aliquota IVA dei giochi. È assurdo e paradossale che l'IVA sui giochi sia minore dell'IVA sul pane e sulla pasta. sottolineando la necessità, indicata nel punto 16), di prevedere una moratoria per le nuove autorizzazioni, in attesa della riorganizzazione e pianificazione dell'intero sistema. Sono tutte questioni che abbiamo condiviso con altri partiti, non solo di maggioranza come il PdL e Scelta Civica; le riteniamo importanti e chiediamo al Governo di condividerle e di portare avanti quanto previsto da questo ordine del giorno.

la controprova è ammessa quando dalle alzate di mano

in questi giorni si sono succedute su giornali e televisioni le dichiarazioni del pentito di camorra Carmine Schiavone. In realtà, non si tratta di nuove rivelazioni, ma di conferme di quanto questi ebbe a dichiarare nel corso degli anni nel processo «Spartacus». Cito una parte dell'intervista più recente, riportata nell'edizione di ieri - 4 settembre - del quotidiano «Latina oggi»,

Cito una parte dell'intervista più recente, riportata nell'edizione di ieri - 4 settembre - del quotidiano «Latina oggi», riguardante lo sversamento di rifiuti tossici in località Borgo Montello, a pochi chilometri dalla mia città, Latina: «Ora ho letto sui giornali che a Latina hanno fatto degli scavi per cercare quei rifiuti, ma hanno scavato da un'altra parte, non quella dove sotterravamo i bidoni, quelli sono nei terreni delle nostre aziende, sempre a ridosso delle discariche, ma da un'altra parte. Dopo aver raccontato tutto alla DDA e alla Commissione parlamentare sulle ecomafie, feci anche diversi sopralluoghi in elicottero insieme a investigatori importanti, e indicai i luoghi esatti dove interravamo i rifiuti chimici. I magistrati volevano che fossero scavati e recuperati, ma la DIA non voleva che quei fusti saltassero fuori. Ho fornito anche i documenti sulla provenienza dei rifiuti, i nomi delle aziende e perfino le targhe dei *camion* che li trasportavano, ma non è successo niente. E hanno secretato tutti i verbali con le mie dichiarazioni rese alle Commissioni parlamentari. Vogliono che la gente muoia in silenzio». Forse era comprensibile mantenere riserbo nel periodo strettamente attinente alle indagini, ma oggi, dopo oltre quindici anni, pretendo di sapere quanto ci sia di vero in queste dichiarazioni. Pretendo di sapere a quali valutazioni di carattere politico, giuridico o sociale si può subordinare il diritto alla salute e all'incolumità stessa dei cittadini. E soprattutto se quanto dichiarato da Schiavone corrispondesse a verità. Pretendo si intervenga urgentemente per evitare ogni ulteriore pericolo per la popolazione residente e per individuare e punire i colpevoli e i responsabili. In caso contrario, la responsabilità di ogni malattia, di ogni vita compromessa ricadrà su questo Stato. Davanti alla vita delle persone non c'è segreto che tenga e anche per questo motivo preannuncio un'interrogazione sul tema, nella sincera speranza che non sia necessario attendere la risposta perché i miei concittadini conoscano quella verità che, semplicemente, è loro diritto.

Signor Presidente, colleghi, cosa ci dà la misura dell'efficacia della nostra azione? Ritengo che i migliori indicatori siano la prosperità del Paese e il senso di affezione dei cittadini verso le istituzioni. Perché ciò avvenga ci vogliono coraggio e inventiva, ma, soprattutto, occorrono la motivazione, il sentirsi cittadini tra i cittadini e capirne i desideri e le paure. Ci sono pezzi del nostro Paese in cui la prosperità non è neanche un ricordo, le istituzioni sono viste come nemiche e le forze dell'ordine - loro malgrado - come repressione e non come protezione. Uno di questi posti è Niscemi, a causa del MUOS. Ho visto la base americana che accoglie il cantiere del MUOS: sta in mezzo ad una riserva naturale, come uno sfregio su un viso bellissimo.

ultimi giorni, mi sono arrivate telefonate, messaggi e richieste di aiuto disperate. Ritirata la revoca delle autorizzazioni da parte del presidente della Regione siciliana, le gru nel cantiere MUOS hanno ricominciato a funzionare. Le donne di Niscemi e le mamme «No MUOS» piangono. Colleghi, questo è un segnale pessimo. Quella gente - la mia, la nostra gente -che ha chiesto il nostro intervento

chiedere alla Marina americana e agli Stati Uniti di andare a costruire il MUOS in un altro posto, lontano dai centri abitati perché, perché, sperando che non sia mai usato in guerra, possiamo quanto meno essere sicuri che non faccia danni in tempo di pace.

Presidente, la invito a trattare un tema molto delicato, che attiene come metodo al rapporto tra il Parlamento e il Governo. Mi riferisco ancora una volta alla vicenda della chiusura dei piccoli tribunali. Si sta rischiando di mettere in crisi il rapporto tra il Parlamento e il Governo perché ci giungono notizie - vorremmo essere informati al riguardo - che il Governo sta prendendo decisioni che di primo acchito, almeno dalle prime informazioni (mi auguro di sbagliare), sono in nettissima contraddizione con le indicazioni più volte sancite con voti espressi dal Parlamento. Le indicazioni che abbiamo fornito erano oggettive, motivate, serie e coerenti con la riforma, in grado di evitare

dalle prime notizie che giungono, sono in netto contrasto con il Parlamento. Anche sul merito, pertanto, è un patatrac. Quindi, invito fortemente la Presidenza a mettere «la schiena diritta» e a fare in modo che le prerogative del Parlamento nel metodo e nel merito siano finalmente rispettate.

però devo rilevare che vi è stato un ritardo della Presidenza

possibile, convocato per riferire in Senato perché finalmente si giochi a carte scoperte per fugare i timori o i sospetti circa i provvedimenti che, come diceva il senatore Caliendo, in queste ore e in questi giorni si stanno centellinando la salvezza (anche se temporanea, a quanto pare) di alcune sezioni distaccate di tribunali e per dare a questa assise una visione chiara di quello che sta succedendo in maniera apparentemente un po' sotterranea o che comunque noi parlamentari non riusciamo a comprendere.

Certamente però il suo richiamo è fondato. Durante i vostri interventi la Presidenza ha già rappresentato al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Patroni Griffi e al sottosegretario alla giustizia Ferri lo sconcerto dell'Aula (che è anche della Presidenza, ricordando l'ordine del giorno approvato in Senato) rispetto a decisioni che dovessero essere assunte non conformi alla volontà del Senato.

si augura che non vengano assunte decisioni nelle prossime ore che non siano in sintonia non solo con i disegni di legge non ancora approvati o discussi, ma con l'ordine del giorno che fu approvato, credo

a tenere conto degli interventi che sono stati svolti a fine seduta affinché non vengano assunte decisioni arbitrarie. Naturalmente, poi il resto è affidato alla dialettica